Onorevoli colleghi, commemorare a 22 anni dalla sua scomparsa Roberto Ruffilli significa rievocare l'altissimo contributo dato al Paese da uno dei maggiori storici e studiosi italiani dello Stato e della politica. Di lui ricordiamo gli approfondimenti sull'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo; sulla trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare attenzione al cambiamento degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria e unita; alla formazione della nostra Costituzione; alle riforme istituzionali. Al suo contributo teorico e, insieme, di pratica politica si può guardare oggi con rinnovata attenzione per l'evidente attualità delle sue proposte e per l'alta visione che le nobilitano, nella grande tradizione del riformismo democratico cristiano. Dopo un percorso di studi e accademico di altissimo prestigio, la Democrazia Cristiana lo volle responsabile del Dipartimento "Stato-Istituzioni" per poi presentarlo, quale proprio candidato, al Senato, ove fu eletto il 20 giugno 1983 e, quindi, il 15 giugno 1987. In entrambe le legislature, egli è componente della Commissione affari costituzionali; tuttavia, è la sua partecipazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, nel biennio 1983‑1985, che consente al suo pensiero riformista di svilupparsi pienamente. Da responsabile del Gruppo democratico cristiano, egli si concentra sul tema della forma di governo. Su questo le sue intuizioni appaiono di straordinaria attualità. Penso, innanzitutto, al punto di partenza di ogni possibile modifica che egli vede nel Parlamento, il quale va a suo giudizio potenziato attraverso un riordino del bicameralismo capace di eliminare le duplicazioni che rallentano il processo decisionale, pur mantenendo l'originaria struttura voluta dal Costituente di organo unitario, ma distinto tra Camera e Senato. E nel Senato egli continua a vedere le irrinunciabili radici della volontà popolare e dell'esercizio della funzione legislativa. La sua visione del Parlamento lo porta a sostenere il rafforzamento della funzione di controllo delle Camere e una maggiore chiarezza - forse oggi la potremmo intendere come separazione di competenza, nella condivisione del potere - tra il Legislativo e L'esecutivo. Più in generale, la lettura strategica delle riforme istituzionali coniuga l'esigenza di governabilità e stabilità con quella della indispensabile partecipazione dell'elettore all'esercizio del potere. Quest'ultimo elemento è per Ruffilli la massima garanzia del principio di uguaglianza e di democraticità. È questa la traccia dossettiana che si scorge nel suo pensiero e si manifesta rileggendo l'insieme degli interventi nella Commissione Bozzi e nel suo studio sulle riforme, dall'eloquente titolo: «Il cittadino come arbitro». al suo lascito intellettuale non si può dimenticare l'altra grande preoccupazione di Roberto Ruffilli, quella sul ruolo insostituibile rivestito dai partiti. Ai partiti deve essere chiesto - questa già allora la sua esplicita convinzione - di indicare, prima della competizione elettorale, la coalizione di governo che, vincendo, andranno a formare, così da avere un sistema nel quale coalizioni politiche alternative si possono alternare alternare alla guida del Paese. È questa la via per far essere i cittadini protagonisti - veri arbitri - nel confermare o cambiare le maggioranze di governo. Egli metteva in guardia contro il rischio di una crescente delegittimazione del nostro sistema democratico. Era un uomo che aveva vissuto nel modo più alto l'insegnamento di Aldo Moro, anche riguardo agli squilibri e alle tensioni della società italiana, ai quali pensava si dovesse far fronte rinsaldando le istituzioni nella coscienza popolare e collettiva, vincendo tutte le forme di protesta, di rifiuto, di separatezza. Proprio in questo straordinario esempio di coinvolgimento dei cittadini, attraverso un progetto riformista di rinnovamento della democrazia, si rinvengono le radici del suo sanguinoso assassinio, perpetrato dalle Brigate rosse. I terroristi vedevano nella sua persona un filo che lo legava ad Aldo Moro, a Ezio Tarantelli e a Vittorio Bachelet. La crudele idea dei terroristi di uccidere coloro che esprimevano con la loro presenza e iniziativa una sintesi tra mondo della cultura e politica, si rivelava un proposito disumano, irrazionale, senza prospettive, certamente, ma che, purtroppo, anche molti anni dopo sarebbe sopravvissuto a quella stagione di sangue e di dolore e avrebbe portato ai delitti di Biagi e di D'Antona. Roberto Ruffilli fu assassinato il 16 aprile 1988, a dieci anni dall'assassinio di Aldo Moro, pochi giorni dopo la formazione del nuovo Governo De Mita, alla cui nascita aveva dato un diretto contributo.

"uno dei migliori quadri politici della DC, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente». Questa era la sua colpa per i terroristi. Onorevoli colleghi, noi oggi commemoriamo Roberto Ruffilli per tanti e profondi insegnamenti che sono sopravvissuti alla sua persona. È questa la prova della grandezza dell'intellettuale e del politico, di cui voglio ricordare una lezione di metodo che credo sia valida ancora oggi per ogni riformista, quale che sia la sua ispirazione culturale o ideale. «Si tratta» - diceva Ruffilli - «di corrispondere alle attese dei cittadini per riforme che eliminino occupazioni abusive dello Stato e della società e che potenzino governabilità dei rami bassi e dei rami alti senza metterne in discussione i rami altissimi: quelli dei principi fondanti della Costituzione. Tutto ciò per ovviare ai fenomeni crescenti di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, bloccando il logoramento delle conquiste della democrazia repubblicana, specie a proposito della partecipazione popolare all'esercizio del potere». Parole che, ancora oggi, ci servono di insegnamento, ci indicano un percorso, sottolineano i compiti e i doveri di una politica degna di questo nome. Signor Presidente, oggi, commemorando Roberto Ruffilli in occasione del del 22° anniversario della sua morte, ricordiamo un uomo politico che poteva contare su una profonda conoscenza delle problematiche del suo tempo; una figura mite e serena. Fu uno studioso, prima ancora che personalità importante del Parlamento italiano. Da analitico, Ruffilli ha sempre sottolineato la funzione insostituibile dei partiti, così come la centralità e il potere decisionale del cittadino. La formazione di storico si confondeva in lui con la passione per la politica, portandolo sempre alla ricerca delle radici profonde delle crisi per meglio comprendere il presente. Animato da questo spirito, si impegnò a fondo nell'analisi dell'ordinamento dell'Italia unita. L'anniversario della sua morte cade in giorni in cui le riforme sono al centro del dibattito politico; ci sarebbe forse stato utile conoscere il suo pensiero, di lui che fu promotore delle riforme istituzionali. A tal proposito, Ruffilli condivideva l'urgenza di semplificare lo svolgersi dei processi decisionali, convinto che ogni innovazione istituzionale dovesse avanzare senza prescindere dalla "complessità" della vita democratica italiana. Quello che Ruffilli riuscì a prevedere e cercò di dimostrare fu che ogni *deficit* democratico si supera muovendo dalla contestuale ridefinizione sia delle forme istituzionali, sia dei diritti e dei doveri propri dell'arbitro della democrazia, cioè del cittadino. Quando venne eletto al Senato della Repubblica, nelle fila della Democrazia cristiana, pose la sua preparazione al servizio dello Stato, lavorando sempre per il perseguimento del "bene comune", un tema oggi di grande attualità: è quel bene comune a cui hanno fatto riferimento il Capo dello Stato e il Santo Padre, richiamando alla responsabilità l'intera classe politica. Mi piacerebbe che ricordarlo in questa sede possa assumere un significato più ampio: vorrei che tornasse alla mente l'esempio di uomo politico Ruffilli divenne una figura scomoda perché fu la dimostrazione vivente che la Democrazia cristiana era attenta ai problemi reali della gente. Contrariamente a quanto le Brigate rosse sostenevano, con lui la Democrazia cristiana dimostrava grande attenzione alla povertà, alle fasce deboli, ai problemi dei lavoratori. Egli lavorò su quello che era un terreno privilegiato dai terroristi, ma che rappresentava anche il suo terreno naturale: cioè il sociale. Non solo: le Brigate rosse temevano anche le capacità mediatrici di Ruffilli. Nella giustificazione farneticante rilasciata nel comunicato firmato dalla stella a cinque punte, egli fu vittima prescelta per la parte attiva avuta parte attiva avuta nel «ricucire tutto l'arco delle forze politiche, comprese le opposizioni istituzionali». A molti giovani il suo nome risulta meno noto rispetto a quello di altre personalità del periodo; Ruffilli fu una persona discreta, che lavorò a lungo nell'ombra, adoperandosi per quel Governo che vide la luce pochi giorni prima della sua morte, cioè il Governo De Mita. Fu un'uccisione brutale, che lasciò la sua Forlì e l'Italia intera senza parole, a dieci anni esatti dall'assassinio di Aldo Moro. Un decennio caratterizzato da ripetuti attacchi terroristici contro magistrati, imprenditori, personalità politiche e sindacali. Furono i famigerati anni di piombo, durante i quali i terroristi, in nome di falsi ideali e di contradditori principi rivoluzionari, fanatici dell'anarchia, non esitavano a colpire illustri personalità della nostra società, ritenute responsabili di ineguaglianze sociali e di asservimento all'imperialismo. Dalla violenza che caratterizzò quel periodo nacque nel popolo italiano un forte sentimento di rifiuto e di condanna di tale ideologia, un sentimento che ha contribuito a rafforzare la nostra democrazia. Oggi viviamo con orrore le reminescenze di quegli anni: nuovi gruppi terroristici, figli di quell'epoca, intenzionati proprio a tornare alle origini, a rilanciare la lotta armata mediante attentati in nome di una prospettiva antimperialista e anticapitalista, riproponendo la sigla delle Brigate della stella a cinque punte. Questo fa capire che non si può abbassare la guardia, ma che è necessario piuttosto intensificare la lotta al terrorismo, sradicando sul nascere i focolai eversivi. Vorrei concludere dicendo che il modo migliore di ricordare il sacrificio di quanti lottarono per un Paese migliore e per una solida democrazia è rafforzare quel cordone ideale che ci vede l'uno a fianco all'altro, al di sopra di qualsiasi ideologia politica, a difendere la democrazia, che costituisce l'identità stessa del nostro Paese, impagabile eredità lasciataci dai nostri padri e che abbiamo il dovere di consegnare intatta ai nostri figli.

Presidente, onorevoli colleghi, il 16 aprile 1988, a dieci anni dall'assassinio di Aldo Moro, le Brigate rosse uccidevano barbaramente a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffìlli. Veniva da una storia personale non facile: figlio, presto orfano, di un operaio di Forlì, la sua formazione se l'era dovuta costruire quasi da solo, nel dopoguerra, unendo alla frequentazione dei circoli cattolici e poi degli stimolanti ambienti milanesi della Università cattolica quella voracità da autodidatta che sarebbe rimasta una sua caratteristica, facendone in età matura un lettore onnivoro. Vogliamo oggi ricordare la sua straordinaria capacità di stabilire terreni di comunicazione con chi militava in differenti ed opposti campi culturali. In questa sua dote pesavano moltissimo la sua onestà intellettuale e la capacità che aveva di ragionare insieme con gli altri. Non era semplice inclinazione al compromesso ideologico, perché anzi nella discussione non mollava, sapeva essere intransigente sino alla polemica. Era, piuttosto, una vocazione alla tolleranza che gli derivava forse dalla consapevolezza della complessità del mondo e dalla certezza, tutta cattolica, della sua strutturale imperfezione. Piuttosto che storico preferiva definirsi «scienziato sociale»: guardava cioè alla sociologia nella chiave di un'antica e mai tradita fedeltà a Max Weber; puntava ad una storia delle organizzazioni che non dimenticasse la dimensione del sociale, aperta all'apprezzamento del mutamento e insieme delle persistenze culturali di lunga durata, disponibile alla comparazione tra casi nazionali differenti. Vinto un concorso a cattedra di storia contemporanea, fu chiamato a Bologna, dove avrebbe poi insegnato sino all'ultimo nella facoltà di scienze politiche. Eletto senatore in un collegio romano, diviene uomo di punta - com'è già stato ricordato - delle riforme costituzionali: paziente ma sfortunato tessitore di una tela riformatrice che purtroppo si romperà troppo presto. Mantenne sempre il suo stile semplice e sereno, di intellettuale discreto, di persona mite e attenta ai problemi e alle posizioni di tutti. L'ampio contributo di Ruffilli allo studio del nostro sistema politico attraverso libri, saggi, pubblicazioni, ma anche articoli di stampa, convinto che ogni uomo abbia il dovere di non estraniarsi dal suo tempo e il dovere di esercitare la responsabilità propria di ogni uomo di cultura, confluiscono nel vasto e attualissimo dibattito sulle riforme istituzionali. Nella sua analisi il Parlamento, presidio delle libertà repubblicane, rimane il punto di partenza e va potenziato attraverso un riordino del bicameralismo, che elimini le inutili e farraginose duplicazioni, ma che mantenga l'originaria struttura voluta dai Padri costituenti di organo unitario distinto, con radice nella volontà popolare e nella funzione legislativa. Esige maggiore chiarezza nel rapporto tra il legislativo e l'esecutivo attribuendo ad ognuno, senza confusione, il ruolo ad essi proprio. L'ideale che lo ispira è quello della democrazia intesa come costruzione continua, rivolta a garantire spazi sempre più ampi di libertà e di partecipazione. Le riforme delle istituzioni devono risolvere i problemi della governabilità e della formazione di maggioranze stabili, ma anche quello di una sempre maggiore democraticità, con la garanzia dell'uguaglianza e con la promozione di una partecipazione reale del cittadino. Per chi come me da giovane, insieme ad altri, ha vissuto gli anni di piombo e il periodo tormentato del '68, l'emozione in quest'Aula è davvero forte. Il terrorismo, allora delle Brigate rosse, oggi internazionale, è la non democrazia. E il costante rinnovamento delle istituzioni e della politica, secondo la lezione che era propria del senatore Ruffilli, è quel comune e concorde lavoro che può estirpare le radici della violenza e assicurare condizioni di convivenza pacifica e laboriosa nella preminente difesa della dignità e della libertà della persona A me interessa oggi in quest'Aula, caro Presidente, rivolgermi alle nuove generazioni, perché questo è il messaggio della giornata. La riflessione attorno a una figura di questo spessore del Novecento ci interroga e interroga il Paese. Allora voglio dire ai giovani che si affacciano al davanzale del terzo millennio che credo che a loro vada la freschezza di questa memoria, capace di suscitare nelle loro coscienze il bagliore di una nuova speranza, l'invito all'impegno civile. Allora io credo, cari colleghi, che quel sacrificio, il sacrificio di quella vita drammaticamente spezzata può essere e farsi seme di libertà.

vorrei ringraziarla in modo sincero per i contenuti della commemorazione che ha reso in quest'Aula, perché li ho trovati pienamente rispondenti alla vicenda umana e politica del senatore Ruffilli e tali anche da riconoscere il giusto valore ad una stagione politica appena abbozzata, quella della seconda metà degli anni Ottanta che, se avesse sortito esito migliore, avrebbe dato a questo Paese un futuro meno drammatico e meno attraversato dalle turbolenze che poi seguirono. Infatti, all'indomani del 16 aprile del 1988, di fronte a quell'assassinio, furono in molti a domandarsi chi fosse la persona divenuta bersaglio di tanta violenza. Le Brigate rosse lo assassinarono brutalmente nella sua casa con una vera e propria esecuzione, facendolo inginocchiare e sparandogli tre colpi alla nuca. Vollero uccidere, anche simbolicamente e dichiaratamente, il lucido intellettuale che sapeva ispirare e animare lo sforzo riformatore che agli inizi degli anni Ottanta caratterizzò l'allora segreteria della Democrazia cristiana. Un libro a lui dedicato, «Roberto Ruffilli: una vita per le riforme», credo che sia il modo più corretto per ricordarlo, nel suo impegno di studioso soprattutto, ma anche di parlamentare e membro di quest'Assemblea dal 1983 e per troppo poco tempo. Roberto Ruffilli ha avuto a cuore, come pochi, la riforma della politica e l'ammodernamento del nostro sistema istituzionale. A lui si deve l'idea del cittadino arbitro, il cittadino cioè che prende nelle proprie mani la scelta di maggioranza che esprimerà il Governo. La follia omicida del terrorismo individuò in lui un obiettivo da abbattere in quanto protagonista di primissimo piano di una stagione che si annunciava di trasformazione e modernizzazione dell'architettura istituzionale legata, imprescindibilmente (perché questa era la cifra politica di Ruffilli), ad una riforma dei partiti: diciamo riforma, non svilimento, perché lo studioso forlivese, che si era formato alla scuola dei più grandi nomi della cultura cattolico-democratica, aveva ben chiara la rilevanza politica e sociale dei partiti, così come prescrive la Costituzione all'articolo 49. Ma gli stessi partiti dovevano cambiare e questo a Ruffilli era ben chiaro. Credo si possa dire, con estrema certezza, che se il processo riformatore al quale lavorava Roberto Ruffilli, non si fosse fermato con la sua tragica scomparsa, la crisi della cosiddetta Prima Repubblica, che ha visto una sorta di «rottura» della continuità istituzionale e democratica, non ci sarebbe stata, poiché avremmo avuto, probabilmente, un processo riformista che avrebbe adattato le nostre istituzioni ad un Paese che stava cambiando, socialmente e politicamente. Oggi, a quasi vent'anni di Seconda Repubblica, noi torniamo a parlare di riforme delle istituzioni in un Paese investito da una condizione di recessione economica gravissima da molti anni, dove ad ogni appuntamento elettorale il disincanto del cittadino verso la classe politica si manifesta nel fortissimo assenteismo elettorale e con un quadro di relazioni istituzionali totalmente sfilacciato, a cui si tenta di rispondere evocando sempre più la suggestione di una democrazia plebiscitaria, piuttosto che articolare la democrazia in termini moderni ed efficienti. Credo quindi che il modo migliore per rendere onore a questo martire della democrazia italiana sia procedere con speditezza, ma anche con oculatezza, lungo la strada tanto evocata delle riforme. Sappiamo tutti, infatti, che taluni dei mali che affliggono il nostro Paese sono dipendenti da un sistema che rende farraginosi i processi decisionali e, nel contempo, sottrae al Parlamento quote di potestà legislativa e di funzione di controllo. Ma se vogliamo trarre un vero insegnamento, o più modestamente, una qualche ispirazione e un senso politico vero dalla memoria di Roberto Ruffilli, dobbiamo intanto ritornare ad affidare al «cittadino» la possibilità di scegliere, non soltanto il capo della maggioranza di Governo e, forse domani, il Capo dello Stato, ma anche e soprattutto i suoi parlamentari, restituendogli lo scettro della sua decisione proprio quando si tratta di indicare colui che lo rappresenterà in queste Aule, decisione che gli è stata sottratta dall'attuale legge elettorale. Questo rappresenterebbe il modo migliore per onorare la testimonianza e l'eredità umana, culturale e politica di Roberto Ruffilli, che resterà una delle intelligenze più nobili della nostra Repubblica.

Grazie, politiche nel 1960 seguirono gli studi presso l'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica, a Milano, dove svolse anche tirocinio di ricercatore. Nel '68, in un periodo difficile della vita universitaria, all'epoca della contestazione, Ruffilli svolse anche l'attività di rettore al Collegio Augustinianum, che lascia nel '70 per volgersi più intensamente agli studi sulle riforme istituzionali.

valenza al suo pensiero politico, che fu coerente con quello di studioso. Gli studi di Ruffilli, infatti, non hanno avuto solo una valenza accademica, ma hanno individuato precise strategie di azione politica. Ai partiti, ad esempio, ha sempre attribuito una funzione insostituibile per la vita democratica. Ad essi, nelle sue teorie e nelle sue proposte politiche, chiese di chiese di scegliere anticipatamente, in sede di competizione elettorale, la coalizione di Governo, tanto da pervenire ad un sistema nel quale le aggregazioni politiche si fossero predeterminate in campagna elettorale e alternate al governo del Paese. Ecco quindi che il cittadino diventava come è diventato: vero arbitro del cambiamento di una maggioranza di Governo, non assegnando ai partiti una delega in bianco che avrebbe rischiato di svuotare i contenuti di un mandato elettorale. È un pensiero degli anni '70 e '80 che riteniamo quanto mai valido un pensiero che nella realtà dei fatti l'attività politica istituzionale ha perseguito e realizzato. Ecco però che probabilmente per questa visione la sua vita fu stroncata dalla mano assassina delle Brigate Rosse, nel 1988. È esplicativa al riguardo

non solamente nella forma istituzionale, ma anche nella competizione, basata su espliciti programmi alternativi, riconoscibili dal cittadino elettore. Parlava anche di un bicameralismo differenziato, del rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, di riforme delle istituzioni che dovevano essere affiancate e sostenute sostenute anche da una riforma che facesse evolvere ruoli e funzioni delle autonomie locali. Ruffilli era consapevole che qualsiasi rinnovamento dell'ordinamento istituzionale non poteva negare il valore alle alle realtà territoriali né l'azione normativa da esse espressa. Per questo, ancora oggi il suo progetto di riforma mantiene una profonda attualità. Ad esso, quindi, è utile richiamarsi nell'affrontare i problemi di un miglior funzionamento delle nostre istituzioni democratiche. Per questo, infine, è opportuno sottolineare l'estrema attualità del messaggio politico di Roberto Ruffilli.

Signor Presidente, ventidue anni fa, il 16 aprile 1988, degli uomini vili, tragicamente convinti che le idee avanzino sulla punta dei fucili, diritto e di storia contemporanea, senatore della Repubblica, per alcuni di noi amico mite, generoso e guascone. Le Brigate rosse, con la stessa mitraglietta Skorpion con cui avevano assassinato Ezio Tarantelli, l'ex sindaco repubblicano di Firenze, Lando Conti, e due giovani agenti di polizia a via Prati di Papa a Roma, Rolando Lanari con modi simili a quelli usati dai carnefici nazifascisti - due colpi alla nuca della vittima inginocchiata - spensero la vita, ma non l'opera di una figura politica luminosa del cattolicesimo democratico e della politica italiana. Oltre la cronaca di quel giorno, che alcuni di noi serbano con dolore nel cuore, credo sia possibile rendergli omaggio seguendo due direzioni di lettura: l'impegno per le riforme istituzionali come servizio al cittadino, al "cittadino-arbitro", come scrisse assieme a Capotosti, e l'opinione sul perché della fredda esecuzione di un uomo di studi, politico sensibile e anche tenace, ma certamente non esercitante una *leadership* esterna così in vista. Le riforme istituzionali, di cui oggi si torna a parlare, con la Commissione Bozzi, di cui ovviamente Ruffilli faceva parte, ebbero una prima fase di impegno e di entusiasmo, in cui sembrava davvero possibile, agli albori della crisi di credibilità dei partiti politici, una riforma condivisa. Come sappiamo non fu così e oggi ci ritroviamo con quesiti simili, in una condizione di relazione peggiorata tra la società civile e la politica. Riferendosi a quel lavoro comune, in un'intervista a pochi giorni dal suo assassinio, Ruffilli disse che vi erano alcuni punti di unione che oggi possono ancora essere considerati un viatico al nostro lavoro: un bicameralismo differenziato ed un rafforzamento delle funzioni di legislazione, di controllo e di indirizzo del Parlamento; un consolidamento della posizione del Presidente dei Consiglio dei ministri; una articolazione del sistema delle fonti che valorizzi la legge parlamentare, il potere normativo del Governo, la potestà legislativa regionale. Inoltre, che fosse puntualizzata la responsabilità del soggetto che determina il governo dell'economia. «Siamo così al di fuori» - disse - «delle grandi semplificazioni (...) ma abbiamo anche bisogno» - e vale anche per l'oggi - «dell'apporto critico di una opinione pubblica che metta i partiti politici di fronte alle proprie responsabilità (...) evitando la scappatoia della ricerca di mitiche riforme globali e perfette». Era chiaro in Ruffilli, insomma, che le riforme servono per favorire scelte politiche a favore di contenuti chiari e condivisibili dei cittadini e non per soddisfare ansie accademiche, oppure per sviare il discorso dalle condizioni di bisogno del Paese. Per questo, colleghi, sarebbe riduttivo dire che Roberto Ruffilli era un «professore prestato alla politica». Lo compresero bene le Brigate rosse - e qui rifletto sulla seconda questione annunciata ebbero la capacità strategica di identificare in Ruffilli colui che stava lavorando sulla parte più ambiziosa del programma del Dicastero De Mita, ovvero il tentativo di offrire a tutto il Parlamento, opposizioni comprese, una chiave di riforma complessiva delle istituzioni. Caro Presidente, questo è un tarlo intellettuale, che lei ha ben indicato nel suo intervento e che non erode solo noi cattolici democratici. Credo sia giusto qui chiederci perché questa scelta scellerata, ma così strategicamente pensata, di Ruffilli. Noi rimanemmo colpiti dalla spietatezza dell'assassinio a confronto della mitezza, anche nei modi, del rispetto per competitori ed avversari, certo, certo, ma anche dalla geometrica potenza di lettura delle Brigate rosse, che conoscevano - lo testimoniano i comunicati di rivendicazione - Ruffilli più dello stesso sistema politico-mediatico. Non era certo la geometrica potenza espressa in altro modo a Via Fani su Aldo Moro e la sua scorta, ma non possiamo non accomunare questa identica capacità di visione strategica con il martirologio cattolico democratico: Aldo Moro al culmine di un passaggio fondamentale per il Paese; l'uccisione di Piersanti Mattarella mentre apre una stagione di confronto nuovo alla Regione siciliana, oppure il ruolo, defilato politicamente ma istituzionalmente fondamentale, di Vittorio Bachelet; infine, la "tempistica" con cui venne ucciso Ruffilli. Nessun complotto, probabilmente, ma forse il semplice, tragico, riconoscimento di una capacità politica di essere al centro dei crocevia della storia. Io guardo al futuro, anche alle riforme istituzionali, come tutti noi, alla riforma della politica e dei contenuti. Ma io continuo a pensare che valga la pena di ricordare persone e politici come Roberto Ruffilli, perché la comunità dei viventi è fatta di coloro che ci sono e di coloro che non ci sono più.

perché non si stenda su di lui, su loro, "il velo fradicio dell'oblio". Non so neppure più il nome del poveretto che ti ha ucciso, ma io ti ricordo, Bobo. Noi ti ricordiamo, Roberto Ruffilli.

come senatrice e come romagnola, io sono onorata e commossa di ricordare oggi in quest'Aula il senatore Roberto Ruffilli. Io ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente e di poter con lui lavorare, come giovane democristiana, nelle sedi di partito di Cesena e di Forlì. Roberto Ruffilli è stato barbaramente ucciso, con una vera e propria esecuzione ad opera delle Brigate rosse, il 16 aprile 1988. Roberto Ruffilli era nato a Forlì, nel 1937, da una famiglia di modeste condizioni. Dalla madre riceve l'esempio di un'adesione semplice e, nel contempo, solida alla fede cristiana. Cresce, quindi, negli ambienti cattolici di una città, Forlì, in cui le contrapposizioni politiche erano particolarmente accese. Come studente, si distingue per i brillanti risultati che lo porteranno, a 23 anni, a laurearsi a pieni voti alla facoltà di scienze politiche dell'Università Cattolica di Milano, dove ricoprirà il ruolo di direttore del Collegio Augustinianum. Gli anni Ottanta vedono l'inizio della sua partecipazione alla vita politica e, nel 1983, egli diventa senatore per la Democrazia Cristiana. Il suo impegno politico è coerente con la sua formazione di studioso e lo porterà ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, soprattutto per quanto attiene al dibattito relativo alle forme istituzionali ed elettorali. Significativo, in questo senso, è il suo impegno all'interno della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la cosiddetta Commissione Bozzi, da cui emerge come la sua formazione di storico si fondasse su un'autentica passione per la politica ispirata alla formula del cittadino come arbitro. Significative, pur nella loro palese incongruenza, sono le parole con cui le stesse Brigate rosse, proprio il 21 aprile 1988, rivendicarono l'attentato: «Sabato 16 aprile un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato». I feroci assassini lo freddarono con tre colpi alla nuca, un sabato pomeriggio di 22 anni fa, e impedirono così a Roberto Ruffilli di vedere i mutamenti che il nostro sistema politico-istituzionale ha avuto fino ad oggi. Ma nella sua terra le sue idee e il suo lavoro sono ancora vivi. Infatti, al suo nome è stata intitolata la facoltà di scienze politiche di Forlì e, per volontà del compianto senatore Leonardo Melandri, altro grande tessitore illuminato della Democrazia Cristiana e dell'università in cui egli ha insegnato è nata la Fondazione Roberto Ruffilli, che promuove iniziative di studio, di ricerca e di formazione in ambito pubblico, con una particolare attenzione per quanto riguarda gli studenti: quegli studenti che lui ha sempre osservato con grande attenzione, che ha cullato, che ha guardato come il virgulto delle nuove società, quegli studenti delle scuole di Forlì e di tutta la Romagna. Ai tanti amici di Roberto Ruffilli (e in terra di Romagna sono rimasti ancora in tantissimi) e alla sua famiglia va un ricordo deferente ed affettuoso. *(Applausi

le riforme istituzionali-costituzionali, le riforme della politica e, dall'altro lato, le riforme strutturali nell'ambito della politica economica e della società italiana. Il motivo politico invece è il seguente, signor Presidente. Presidente. Cari colleghi, ci sono due modi per uccidere una persona: il primo modo è quello cruento e vigliacco. Le Brigate rosse andarono il sabato mattina a casa di Roberto Ruffilli: non lo trovarono, perché era a pranzo della zia (dove notoriamente si recava il Aspettarono il suo rientro, alle tre del pomeriggio, e lo uccisero nel silenzio della sua casa suonando il campanello e bussando alla porta. Questo è il modo vigliacco con cui le Brigate rosse hanno ucciso Roberto Ruffilli e il modo acuto con cui lo hanno mirato,

impegnarci tutti per evitare la seconda forma di uccisione delle idee, magari non rispondendo a quello che ci dice ancora Roberto Ruffilli in tema di responsabilità della politica sulle riforme istituzionali e sulle grandi riforme economiche e sociali di questo Paese, magari pensando di soffocare le voci libere e le idee chiare che ancora oggi ci sono nel nostro Paese. Spero, inoltre (ma ne sono certo), che in queste Aule si cada nella tentazione di soffocare quelle idee sommergendole di oblio e non aprendo il dibattito sui grandi temi del Paese. Questa è la responsabilità comune che abbiamo nel ricordare la vivezza delle idee di Bobo Ruffilli,

Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura alla Camera dei deputati senza modificazioni, reca il Memorandum d'intesa tra Italia e Indonesia concernente l'apertura dell'ufficio denominato *Indonesian Trade Promotion Center*, fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. Tale atto consentirà una maggiore cooperazione economica e commerciale, ampliando le relazioni bilaterali tra i due Paesi, tenendo conto che l'Indonesia riveste una notevole importanza sul piano commerciale sia per numero di abitanti che per tasso di sviluppo. La quota italiana nel mercato indonesiano

Con l'articolo 1 si stabilisce l'apertura a Milano dell'ufficio *Indonesian Trade Promotion Center* in base al principio di reciprocità, l'eventuale istituzione di un centro di promozione commerciale in una città indonesiana a scelta del Governo italiano, per cui sarà comunque necessario un ulteriore provvedimento legislativo *ad hoc*,

nella pubblicizzazione ed introduzione in Italia di prodotti di industrie indonesiane, nell'assistenza alle missioni commerciali da e per l'Indonesia, nello scambio di informazioni utili al miglioramento del commercio indonesiano, nella conduzione di ricerche e studi, nell'agevolazione della cooperazione tecnica, incluso il trasferimento di tecnologia concernente il commercio.

ma avrà l'assistenza del Governo italiano per l'ottenimento dei visti appropriati per i soggetti che non sono cittadini italiani e residenti permanenti in Italia.

territorio italiano, gli eventuali abusi connessi con le facilitazioni derivanti dall'accordo in esame. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum si compone di tre articoli, il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione introduttiva al disegno di legge assicura che l'attuazione dell'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, come precisato nel parere reso dalla 5a Commissione, l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in altra città indonesiana, previsto come eventualità dall'articolo 1 dell'accordo, potrà avvenire solo con l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Presidente, intendo sottolineare solamente come il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi si inserisce in un contesto di forte rilancio del dialogo politico tra Italia ed Indonesia, culminato il 4 marzo 2009 con la visita del Ministro degli esteri indonesiano a Roma in occasione della conferenza internazionale «Unità nella diversità. Il modello indonesiano per una società del convivere», organizzata dal Ministero degli affari esteri con la comunità di Sant'Egidio.

di sviluppo economica-sociale e soprattutto come modello di convivenza interculturale e religiosa. Il Governo condivide tutte le osservazioni che il relatore ha fatto anche sull'urgenza di procedere all'istituzione

diversa da Jakarta verrà disposta con apposito provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri».

Il mio intervento sarà molto breve: il Memorandum consente la formalizzazione delle aspettative verso l'apertura di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica indonesiana, inserendosi nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche di carattere bilaterale. Serve cioè

che il Memorandum serve a organizzare, coordinare e promuovere una serie di occasioni di carattere economico e commerciale soprattutto per le imprese che sono impegnate nell'*export* e nei rapporti internazionali.

il commercio estero (ICE) a Jakarta, il quale, oltretutto, sta svolgendo un lavoro positivo e apprezzato sia da parte delle nostre imprese che da parte dei partner indonesiani, promuovendo gli interessi compositi della nostra economia, delle nostre piccole e medie imprese e del nostro *made in Italy*. Come sottolineato anche dai colleghi alla Camera, vorrei dunque suggerire al Governo di sfruttare la reciprocità non per aprire un nuovo ufficio, rischiando di duplicare le strutture e confondere le competenze, ma per potenziare l'ufficio ICE già presente in Indonesia, che svolge un egregio lavoro. Questa seconda ipotesi permetterebbe anche di ovviare ad un problema che presenta il Memorandum d'intesa, ossia la mancanza di copertura economica, poiché tale soluzione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per il bilancio pubblico. Altra questione su cui chiedo al Governo d'intervenire d'intervenire riguarda in che modo e in che misura il Governo abbia qualificato e quantificato l'entità della reciprocità di carattere commerciale tra Indonesia e Italia. Mi sembrano prerogative fondamentali, laddove si mettono in campo elementi così forti, che non possono essere assolutamente lasciati al caso, ma debbono essere monitorati partendo da dati certi. L'Indonesia, infatti, con i suoi 250 milioni di abitanti e una forte prospettiva di sviluppo, che in questi ultimi anni ha visto una crescita vertiginosa in termini economici e demografici, rappresenta un'opportunità per le imprese italiane e anche per il nostro Governo, che grazie alle relazioni economiche può contribuire allo sviluppo democratico del Paese, quale solo dopo una dura dittatura è riuscito a trovare una fase di pace e di stabilità. Per questi aspetti di carattere positivo, siamo propensi a favorire il provvedimento in esame mi auguro che il tempo perso in questi anni (in cui le imprese italiane sono andate più avanti rispetto alle istituzioni del nostro Paese nella creazione di rapporti e sinergie con il sistema indonesiano) possa essere recuperato attraverso la definitiva approvazione dello stesso Memorandum

della politica estera italiana, al di là dei Governi che momentaneamente ne hanno la responsabilità. Quindi è un atto significativo, poiché ha questo valore. La terza valutazione che

per tanto tempo ha richiesto una politica protezionistica a difesa della nostra economia, è toccato il compito di essere relatore di un provvedimento che invece va

Signor Presidente, ascoltate le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, il Gruppo del Popolo della Libertà le condivide ed esprime voto favorevole sul provvedimento in esame.

Colleghi, proprio non ci siamo. Volete che si sospenda la seduta? Sono argomenti tali che non è normale che si svolgano così. Io mi rifiuto di svolgerli così. Quindi, prego i colleghi di lasciare libero l'emiciclo, poi vediamo se si riesce ad andare avanti. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deliberato, all'unanimità, di proporre a) negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria con il documento in titolo in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007; b) restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire. intervengo soltanto per chiedere che tutta la vicenda sia rimessa nuovamente all'esame della Giunta, in considerazione anche delle recenti pronunce della Corte costituzionale, che con

conclusione diversa da quella rassegnata attualmente dalla Giunta stessa e quindi con la possibilità di negare complessivamente l'utilizzo delle intercettazioni. Naturalmente, questa determinazione dovrà però essere assunta dalla Giunta e quindi dovrà esserci un approfondimento alla luce appunto delle due ordinanze della Corte costituzionale. Pertanto, Presidente, chiederei che la questione sia rimessa nuovamente alla Giunta delle elezioni e

Signor Presidente, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori esprime condivisione su questa richiesta, oltretutto in considerazione del fatto che nella trattazione che si è già svolta su questa vicenda si era fatto riferimento proprio alla opportunità di attendere queste pronunzie della Corte costituzionale. Poiché la relazione presentata e proposta all'Aula

rimetto alla relazione scritta. Si tratta di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore all'epoca dei fatti Raffaele Iannuzzi e, come lei ricordava prima, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato.

Presidente, come i colleghi potranno leggere nella relazione che è stata distribuita, prima della proposta di delibera si afferma che: «La Giunta ha quindi respinto la proposta della senatrice Adamo di non concedere l'insindacabilità nella seduta del 13 aprile 2010, è stato conferito al senatore Balboni l'incarico di riferire in Assemblea». Non è la prima volta - credo che tutti i colleghi ormai abbiano visto il susseguirsi di questi atti che si riferiscono al senatore Iannuzzi

quali motivazioni diverse ci hanno guidato. Lo stesso relatore, nella sua relazione, esplicitamente richiama l'opinione della maggioranza della Giunta sull'opportunità di difendersi di fronte all'interpretazione della Corte espressa in modo autorevolissimo con più sentenze, base alle quali ci troviamo quasi sempre sconfitti nella difesa che il Senato fa quando la Corte impugna i nostri deliberati su queste materie.

l'attività svolta come parlamentare, che è coperta da tutela costituzionale, e le opinioni espresse in altra forma, per così dire

diritto all'applicazione dell'articolo 68. Si va anche oltre quando ci si richiama all'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista e, più in generale, l'attività politica *tout court*, per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata come parte della più ampia attività di politico, ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale. I colleghi della maggioranza, nel proporre a quest'Aula di concedere l'insindacabilità relativamente

se incorreranno in qualche infortunio sul lavoro, non potranno avvalersi degli articoli che riguardano le immunità parlamentari. Ma i giornalisti

a furore di popolo, fra un po' ci porteranno via quest'ultima nostra competenza, quella di decidere noi stessi su tali questioni, per affidarla ad un altro organismo, considerato che noi dovremmo dimostrare ogni volta di sapere entrare nel merito. Noi ci sforziamo; colleghi possono essere testimoni che in alcuni casi abbiamo detto: sì, effettivamente qui non ci sono elementi e occorre assolutamente ribadire l'insindacabilità; in altri invece - come in questi - non ci sono affatto elementi che possano supportare la vostra richiesta di insindacabilità. quindi un appello per il futuro, al di là di questo caso, perché ogni nostra azione crea precedente, al fine di votare contro il parere espresso dal relatore per le ragioni che ho detto.

in una fase in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni e cittadini e politica non è dei migliori. Credo che questo preoccupi tutti, ossia il distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni, l'opinione negativa da parte dei cittadini. Queste interpretazioni avvalorano l'idea di una casta, cioè di qualcuno che usa quella che era una difesa

Tutte le Costituzioni moderne, come la nostra, che escono da dittature, introducono questi principi per difendere la libertà dei deputati, dei parlamentari, dei rappresentanti del popolo da pressioni dell'Esecutivo, di chi controlla la polizia e gli organi repressivi dello Stato. Quindi siamo ampiamente fuori. In questo modo avalliamo l'idea che un deputato o un senatore possa dire qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto, senza pagarne mai le conseguenze, a differenza non solo di tutti i cittadini, ma dei nostri colleghi consiglieri regionali, di un sindaco, di chi senza queste coperture risponde di quello che fa e di quello che dice. Noi dovremmo sentire questa responsabilità, anche con il nostro voto, di dare dei segnali che io credo il nostro Paese

dal 1992, ossia da quando è operativo il nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, vicende come questa hanno dato luogo a circa 1.200 processi in ordine al conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Di questi 1.200 procedimenti, oltre il 90

Il vero conflitto a questo punto diventa tra la giurisprudenza parlamentare e la Corte costituzionale,

esposta negli atti e nelle sentenze, di grande chiarezza e puntualità. Lo stesso relatore nel documento che oggi si propone all'Aula auspica un salto interpretativo della giurisprudenza costituzionale volto a ritenere sussistente il nesso funzionale in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione, ossia sempre.

a tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino con la sua comunicazione: questo è l'auspicio.

a ritenere insindacabili le dichiarazioni: mi sembra un salto logico e giuridico notevole. Augurarsi l'auspicio di un salto interpretativo potrebbe anche avvenire in direzione della giurisprudenza parlamentare: se dopo 18 anni continuano a darci torto, sarebbe forse il caso che il salto interpretativo lo mettesse in atto questa Assemblea e quella della Camera dei deputati. Questa ostinazione nel voler perdere i giudizi, nel farci dire di no in oltre mille occasioni è qualcosa veramente il masochismo. In questa vicenda il nostro ex collega Iannuzzi si è difeso in Commissione assumendo di essere divenuto senatore proprio perché in tal modo avrebbe acquistato la libertà di dire qualunque cosa.

strumentale alla sua attività principale che è quella di poter esprimere le sue idee, anche offendendo. In questo modo,

(perché questo scrisse il senatore Iannuzzi), attribuendogli quindi una condotta idonea ad indurre alla disperazione un uomo sino al gesto estremo del suicidio, è un'opinione: ma questo è un fatto, non è un'opinione.

avesse un intento diffamatorio, evidenziando invece come lo stesso fosse esclusivamente volto a richiamare l'attenzione su alcune indubbie anomalie che avevano contraddistinto la gestione dei pentiti in relazione ad un processo di rilievo, come quello che vedeva imputato l'onorevole Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli». Ma questa sua attività, in ordine alle pretese anomalie nella gestione dei collaboratori di giustizia, non c'entra proprio nulla con ciò che ha scritto: ciò che è stato scritto non riguardava le anomalie nella gestione dei pentiti, ma che i magistrati avessero indotto un uomo a suicidarsi, che è cosa diversa. È stata quindi anche una difesa abbastanza maldestra, che vorrebbe far refluire nell'attività parlamentare di attenzione al fenomeno dei collaboratori di giustizia e alla gestione di questi ultimi un'attività che è diversa,

il momento per il Senato, proprio al fine di rispettare e chiedere una puntuale applicazione della prerogativa che attiene alle nostre funzioni, di cambiare giurisprudenza. Forse uno spiraglio si sta aprendo. Il caso vuole che nell'altro ramo del Parlamento in una vicenda analoga sia incappato un parlamentare dell'Italia dei Valori e la Giunta stia cambiando opinione, nel senso di ritenere che le offese devono essere contenute in atti tipici, quindi non anche in un'attività collaterale della vita politica. Probabilmente siamo ad una svolta storica, epocale. Dopo 18 anni, grazie alle offese che l'onorevole Zazzera avrebbe pronunziato in danno dell'onorevole Mantovano, la giurisprudenza parlamentare cambierà indirizzo. Quindi, non è la Costituzione che deve cambiare indirizzo, ma è la Camera che sta riflettendo su 18 anni di cattiva interpretazione dell'articolo 68. Cerchiamo di essere noi questa volta i primi della classe. Non facciamoci dare lezioni di diritto parlamentare dalla Camera. Rivendichiamo all'Aula sovrana della più alta Camera del nostro Paese questa nostra prerogativa: che sia il Senato per primo a dare questa nuova interpretazione in coerenza con l'articolo 68

ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 22 luglio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale pendente nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2010, n. 130, depositata in cancelleria il successivo 8 aprile e notificata al Senato il 16 aprile 2010. Nella seduta del 20 aprile 2010, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto. La Giunta ha, inoltre, manifestato il proprio avviso favorevole a che il Senato sia rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non

indirettamente anche questo provvedimento si collega al tema generale che era stato da me sollevato, ossia la difesa nelle aule della Corte costituzionale

e paghiamo un costo notevolissimo, in quanto ci si rivolge al libero Foro.

si operasse una scelta nella direzione del risparmio, ossia

che l'Avvocatura generale dello Stato ha manifestato perplessità in ordine alla sua legittimazione ad assumere la difesa

fa, il presidente del Senato, mi pare, se non ricordo male, decise di investire della questione alcuni consulenti accreditati che avessero potuto superare, in positivo o in negativo, il ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato. Abbiamo, peraltro, un precedente recente proprio in una vicenda riguardante un conflitto di attribuizione che contrapponeva il Senato

il Senato si è costituito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento deciso con ordinanza n. 163 del 18-22 maggio 2009. Un anno fa le perplessità erano state fugate

dettato a verbale il profilo attinente l'eventuale non legittimazione ad assumere la difesa del Senato. Essendo stata posta la questione, la Corte costituzionale ha ritenuto implicitamente, perché nel provvedimento non risulta, la legittimazione ad assumere la difesa, tanto è che l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per difendere il Senato. Allora, noi insistiamo, nel prendere questa decisione,

e nelle future che sicuramente si verificheranno, venga affidato all'Avvocatura dello Stato, così da risparmiare il denaro dei cittadini. costo incide sì sul bilancio del Senato, ma si tratta di soldi dei cittadini. Qualora si ritenesse di dare la massima attenzione alla perplessità dell'Avvocato generale avvocato Fiumara, in ordine alla legittimazione, noi insistiamo perché venga sollecitata dalla Presidenza del Senato una consulenza per dirimere

Presidente, colleghi senatori, se noi decidiamo che il Senato si costituisca in giudizio davanti alla Corte costituzionale su questa causa, allora

che questi non avesse invocato l'insindacabilità parlamentare, che non c'è, e avesse accettato un giudizio nel avrebbe potuto difendersi come un normale cittadino. Con la specificità della sua attività politica e degli strumenti che l'attività politica mette a disposizione di tutti noi,

alla costituzione in giudizio per una causa che il Senato potrebbe evitare di perdere in maniera conclamata. Se, tuttavia, la maggioranza ritenesse di dover andare avanti esponendo il Senato ad una ennesima brutta figura riteniamo che si possa sostenere la legittimità della delibera del Senato impugnata in sede di conflitto di attribuzione, mediante gli uffici e la rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. Oltre

testimoniato dall'ordinanza del 22 maggio 2009 nella quale la Corte costituzionale dà atto della costituzione in giudizio del Senato mediante l'Avvocatura dello Stato. Certo, è un giudizio che si interrompe in una inammissibilità del ricorso, ma una volta che il Senato è rappresentato tramite l'Avvocatura dello Stato lo è sia per i profili discussi di procedibilità, sia per quelli di merito.

riflessioni. Vorrei insistere sul punto, non per restare legato ad un convincimento, ma perché ce ne siamo ulteriormente convinti, e ribadire, a nome del Popolo della Libertà, la nostra posizione:

il senatore Izzo aveva suggerito di rivolgere in subordine una raccomandazione al Presidente del Senato secondo la quale, se non avesse avuto esito positivo la

dalle parti della maggioranza su questo punto, voglio allora fare io una raccomandazione al Presidente del Senato, che vale quanto quella del senatore Izzo: il Presidente del Senato consideri l'eventuale disponibilità dei senatori avvocati presenti in quest'Aula, che sono tanti, a rappresentare gratuitamente le nostre posizioni davanti alla Corte costituzionale.